recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)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

Senatori, desidero rivolgere un commosso pensiero di vicinanza e cordoglio ai familiari, ai colleghi e agli amici dell'onorevole Guglielmo Epifani. Sindacalista, politico, uomo delle istituzioni, Guglielmo Epifani è stato una delle figure più autorevoli della Sinistra democratica della nostra epoca. Intellettuale colto e raffinato, si era laureato in filosofia con una tesi su Anna Kuliscioff, fondatrice e tra i principali esponenti del Partito Socialista Italiano. Un'idea, quella socialista, a cui Guglielmo Epifani è sempre rimasto fedele e che ha ispirato ogni importante tappa della sua vita, a cominciare dall'impegno sindacale, vissuto sempre in prima linea all'interno della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL). Un impegno instancabile, fatto di dedizione appassionata e sincera attenzione alle esigenze dei lavoratori. Doti che lo portarono rapidamente ad assumere ruoli sempre più importanti nella segreteria confederale della CGIL e a diventarne, nel 2002, segretario generale. Alla guida del primo sindacato italiano Guglielmo Epifani è stato, per tanti anni, voce forte e coraggiosa dei diritti dei lavoratori. Un sindacalista dialogante ma combattivo, gentile ma tenace e determinato. Un innovatore, sostenitore di riforme anche radicali nel mondo del lavoro un forte promotore dell'affermazione delle donne ai vertici del mondo sindacale. Il suo era un sindacalismo riflessivo e riformista, teso alla ostinata ricerca di una mediazione che potesse unire, attraverso il confronto costruttivo, le posizioni anche più divergenti e contrapposte. Valori che hanno caratterizzato anche il suo impegno parlamentare, iniziato nel 2013 con l'elezione alla Camera dei deputati tra le fila del Partito Democratico, di cui è stato anche segretario reggente, e proseguito in questa legislatura, sempre alla Camera, come esponente del Gruppo parlamentare di Liberi e Uguali. Politico di straordinario spessore etico e umano, Guglielmo Epifani ha saputo interpretare,

seppe conquistare la stima e l'ammirazione di tutti per l'imparzialità, il fermo rispetto delle istituzioni, grandi competenze tecniche e costante attenzione alle istanze di ogni parte politica. La notizia della sua scomparsa è stata motivo di profondo dolore. Con Guglielmo Epifani la politica italiana resta orfana di un galantuomo onesto e leale, di un intelligente protagonista di tante battaglie ai tavoli della concertazione, nelle piazze e nell'Aula del Parlamento. Un *leader* autentico e carismatico, che ha fatto della partecipazione democratica il tratto distintivo del suo impegno sociale accanto ai lavoratori. In ricordo di Guglielmo Epifani invito, pertanto, l'Aula del Senato ad osservare un minuto di commosso silenzio.

ho conosciuto bene Guglielmo. Molti anni fa lo chiamavamo il compagno Ford. Non Henry Ford, però, bensì Harrison Ford. Questo perché era intellettualmente molto preparato. assomigliava più a Bruno Trentin che non a Di Vittorio, era sempre quello in cravatta ed era di una certa raffinatezza. Per cui, rappresentava una CGIL con la quale noi eravamo molto in sintonia. È stato un riformista intransigente. Intransigente perché ha mantenuto un filo nella condotta della sua vita e, sebbene abbia compiuto scelte via via diverse, è rimasto sempre molto leale rispetto alla sua tradizione iniziale. Mi fa piacere che oggi tra i banchi del Governo sieda un caro e vecchio amico, Roberto Speranza,

di stravolgere il mondo e l'Europa, quindi una sorta di Italia felice. Guglielmo guida anche la parte finale di questo percorso, che vede la crisi esplodere negli Stati Uniti nel 2007-2008 e il terremoto terribile de L'Aquila.

ultima esperienza da sindacalista, alla sicurezza nel mondo del lavoro. Si trattava di una questione che aveva intuito e che, purtroppo, gli aveva dato ragione (dico purtroppo perché gli incidenti nel mondo del lavoro in Italia non sono affatto diminuiti). Un abbraccio forte a Guglielmo.

Signor Presidente, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia desidero associarmi sinceramente alle sue parole di cordoglio

Studi classici e laurea in filosofia - lei lo ha ricordato poco fa - con una tesi su Anna Kuliscioff, fondatrice del Partito dei lavoratori italiani, poi

della febbre puerperale e lottò per il suffragio universale, anche se poi non ebbe successo. Credo che da questi studi Guglielmo Epifani abbia fin da giovane deciso da che parte stare: dalla parte dei lavoratori e della giustizia sociale. Questa è stata la cifra del suo impegno di una vita intera. Certo, noi molte volte non abbiamo condiviso le sue idee, le sue opinioni, la parte dalla quale si è schierato e per la quale ha lealmente, con grande sincerità e grande pragmatismo, sempre combattuto. È stato quindi per noi un avversario da rispettare, le cui idee meritavano sempre un confronto, un approfondimento e una sfida per noi che avevamo una visione diversa dalla sua. Questa è la nobiltà della politica che deve sempre avere come punto di riferimento il bene comune. Ecco, Guglielmo Epifani, da avversario, ha contribuito nella dialettica politica al bene comune, alla crescita della nostra società e soprattutto alla crescita dei diritti dei più deboli e dei lavoratori, testimoniando, spesso con scelte che non erano in linea con la sua parte politica, la sua sincerità e la sua onestà intellettuale. Per queste ragioni, Presidente, colleghi, amici di quest'Aula, noi ci associamo sinceramente e profondamente al cordoglio perché non è soltanto una parte politica che ha perso un suo *leader*, ma sono la politica intera e l'Italia la politica intera e l'Italia intera ad aver perso un esponente di cui ci sarebbe stato ancora tanto bisogno in questi momenti così difficili. La sua competenza in materia economica era infatti certamente una competenza utile ed essa, accompagnata al suo equilibrio e al suo pragmatismo, poteva certamente ancora dare frutti importanti per il popolo italiano in questo momento così difficile. *(Applausi)*.

il giorno in cui è scomparso il caro Guglielmo Epifani ero alla sede del partito, c'erano il segretario del nostro partito Enrico Letta e altri membri della segreteria e dei sindacati. Eravamo al tavolo con loro e la notizia ce l'ha data proprio Maurizio Landini. Quel momento è stato per noi l'immagine di tutto quello che aveva rappresentato il mondo di Guglielmo Epifani; il sindacato

in un momento estremamente delicato, era stata affidata a lui anche per le sue caratteristiche: grande integrità,

non si è mai isolato. Come ha ricordato il presidente Mattarella nel suo messaggio di cordoglio, Epifani aveva una visione riformista sempre attenta in tutti gli ambiti, dal sindacato alla politica, rispetto agli interessi dei lavoratori. È stato altresì rammentato nel momento del ricordo civile che uno dei suoi ultimi interventi pubblici è stato proprio a fianco dei lavoratori della Whirlpool, chiedendo al Governo di metterci cuore e risorse. Per lui infatti valevano sempre le parole che aveva ribadito più volte: occorre ridare al lavoro quel senso pieno di diritti, responsabilità e valori. Ha provato a farlo sempre nella sua storia di sindacalista e politico con una lealtà e una passione civile che tutti, avversari compresi, gli hanno sempre riconosciuto. C'è anche una parte del suo impegno giovanile che mi piace ricordare, nei confronti dei ragazzi più fragili e delle famiglie povere. Per i primi infatti faceva ripetizioni gratuite, per i secondi assistenza agli anziani; una empatia e una generosità che raccontano tanto dell'uomo e delle ragioni per cui in tanti ne sentiamo già la mancanza. Non aveva bisogno di farsi notare, di mostrare i muscoli; voleva essere utile e desiderava ottenere degli obiettivi senza rompere. Mi ha molto colpito una frase con cui Sergio Soave ha commentato la sua storia su "Il Foglio": Epifani voleva convincere, non vincere. Quindi era un vincere con, tenendo insieme proprio nel nome di un'unità, perché, quando si vince insieme, si è più forti. «Tutto dipende dalla salute e dalla sicurezza delle persone: lo stato del presente, la possibilità di programmare il futuro, gli interessi economici, la propria dignità, la propria libertà, il proprio lavoro, il sistema degli affetti di relazione». Lo diceva Epifani in occasione del *question time* con il *premier* Mario Draghi il 12 maggio scorso; un intervento in cui chiedeva al *Premier* di aiutare tutti di aiutare tutti noi a vincere questa battaglia culturale e questa sfida di consapevolezza, perché è uno dei sintomi della civiltà e della democrazia del lavoro di un Paese. Lo voglio ricordare con le parole con cui lui ha ricordato Massimo D'Antona. Sono quelle che mi vengono davvero in mente per commemorarlo in quest'Aula, per commemorare la sua grandezza: «Resta la memoria, ma, ancora più della memoria, deve restare (...) il buon esempio che ha dato al nostro Paese, alle istituzioni e alla comunità». Tutta la nostra vicinanza alla famiglia, al fratello e agli amici di LeU e anche di Articolo

Signor Presidente, è con difficoltà e commozione che prendo la parola per ricordare Guglielmo Epifani, una persona che è stata per me un amico; per il mondo del lavoro, per il sindacato e per la sinistra un riferimento irrinunciabile. Anche da qui voglio mandare un abbraccio alla moglie Giusi, al fratello e a tutti i familiari. Dalle tante testimonianze su di lui in questi giorni sono emerse le qualità che lo hanno contraddistinto, da parte degli avversari, dei colleghi e dei compagni. Giustamente gli hanno riconosciuto lo spessore culturale, intellettuale, politico e morale. Sono caratteristiche difficili da trovare insieme in una persona ed erano quelle che hanno fatto di lui un grande *leader* sindacale e politico. Ecco, un *leader*, l'idea giusta del *leader*. La vita di Epifani è stata dedicata alla causa del lavoro, fino alla fine; il suo ultimo atto politico è stato quello di trovarsi insieme agli operai della Whirlpool. Inutile ripercorrere il suo *curriculum*, che tutti conosciamo: socialista, riformista, sindacalista, segretario della CGIL, deputato e segretario del PD, poi l'impegno in Articolo Uno e nella lista di LeU, con la quale fu eletto alla Camera dei deputati. Per Guglielmo il socialismo è sempre stato un punto di riferimento fondamentale, non un elemento consegnato al passato, non un elemento consegnato a una storia finita, ma un sistema di valori e di idee profondamente radicato nel suo modo di pensare e di agire. Queste le parole con le quali ha ricordato il centenario della CGIL nel 2006: «Non abbiamo vissuto e speso questa storia per tornare alle disuguaglianze del tempo delle origini. (...) Lavoreremo perché il futuro abbia il cuore e la forza di questa storia, che è la storia del Paese, rinnovandola e riformandola, accettando le sfide, come sempre abbiamo fatto». Questo è il punto centrale. Il mondo cambia e cambiano le condizioni di lavoro, di produzione, ma ciò che rimane fondamentale è la lotta alle ingiustizie, per affermare i diritti, per affermare il valore del lavoro prima di tutto come idea di dignità. Guglielmo sapeva da che parte stare e sapeva starci anche quando non era comodo. Questo è il vero significato della parola «riformista», che non è un sinonimo di moderatismo; anzi, per essere riformisti bisogna sapere essere radicali. Riformismo è la capacità di calare nella realtà le idee di emancipazione degli esclusi, stare dalla parte degli emarginati, vedere il mondo con i loro occhi. Epifani era un riformista perché sapeva da che parte stare. *(Applausi).* La gentilezza e la correttezza che lo caratterizzavano erano unite a una convinzione nei propri ideali, tali da renderlo sempre disponibile al dialogo, ma fermo, determinato nei propri convincimenti; di quella fermezza sana che unisce il senso della misura e la radicalità. Una fermezza e una determinazione che gli hanno permesso di non essere mai conservatore. Aveva ben presente le grandi trasformazioni della nostra società, a partire dalla frammentazione del mondo del lavoro, ed era consapevole che alla sinistra di Governo, per svolgere una funzione per il Paese, spetta il compito difficile di interpretare il cambiamento, ritrovando la capacità di rappresentare, di guardare avanti senza mai rinunciare alla giustizia sociale. Era un uomo delle istituzioni che ha creduto sempre, fino in fondo, al valore della democrazia e al rispetto dei suoi luoghi e delle sue forme, comprendendo che, senza di queste, la democrazia è una parola vuota. Era razionale e appassionato del merito, avversario della disintermediazione, delle scorciatoie comunicative, della demagogia. Colleghe e colleghi, prima di concludere voglio sottolineare la sua attenzione alle disuguaglianze: quelle sociali, territoriali, di genere. Non era un uomo del Sud, ma la sua sensibilità e attenzione verso il Mezzogiorno erano l'elemento centrale

sembra sempre più povero da un punto di vista umano, un grande vuoto che non potremo mai colmare. Il Parlamento e il Paese perdono un uomo delle istituzioni, un democratico, per i lavoratori un *leader*, per la sinistra, per i socialisti, un compagno. Il sentimento è ora di ringraziamento a Guglielmo per ciò che ha fatto per il Paese, per i lavoratori, per tutte le compagne e i compagni nella lotta per una società più giusta. L'impegno che dobbiamo prenderci è di provare a essere alla sua altezza.

chi ha conosciuto Guglielmo Epifani, o semplicemente ha avuto modo di ascoltarlo, ha capito che era soprattutto una persona perbene. Un uomo che, in qualunque compito si sia cimentato, ha dimostrato una grande coerenza di idee e di propositi, e la coerenza è sempre stata supportata da una grande preparazione. Non è mai accaduto di sentire parlare Guglielmo Epifani di un argomento di cui non avesse cognizione. Questo è il ricordo che abbiamo noi parlamentari, ma anche quello dei cittadini comuni che lo hanno conosciuto attraverso i notiziari o le trasmissioni televisive. Un altro tratto che lo ha caratterizzato è stato la capacità di confrontarsi ascoltando le idee degli altri, senza contrapposizioni sterili, ma sempre in modo costruttivo. La sua provenienza dal mondo sindacale e la sua militanza politica in un sindacato prettamente di sinistra ne ha fatto certamente uno degli uomini migliori di quella parte politica, ovviamente trattava le questioni del mondo del lavoro con grande competenza, che non sempre riuscivamo a condividere, ma di cui capivamo bene le ragioni e apprezzavamo il modo fermo ma pacato di difenderle.

si condividono nemmeno idee e programmi, ma il confronto vero, leale, costruttivo aiuta a crescere, soprattutto se di fronte si ha avuto una persona come Guglielmo Epifani. Difetti e differenze, infatti, si conoscono solo grazie a chi è in grado, educatamente, di farle conoscere. Così si cresce ed Epifani, con la sua storia e le sue battaglie, ci ha aiutato a crescere, a capire e a collaborare. Portare in piazza quasi un milione di persone ne dimostra anche un forte e costruttivo carisma. È stato un uomo che, per il bene della collettività e senza critica, ha sempre affrontato scelte difficili e momenti sindacali complessi. È vero: il sindacato perde un uomo colto e deciso. Epifani sapeva che il suo mondo rappresenta non l'imprenditore, ma il lavoratore, ma, da uomo corretto e non ipocrita, lavorava non per il consenso ma per il bene dei suoi lavoratori. Di Epifani rimarrà un ricordo incancellabile di uomo gentile e mancherà anche a chi non la pensava come lui. Dalla Lega un sincero cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Signor Presidente, colleghi, a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle mi unisco al dolore per la scomparsa di Guglielmo Epifani ed esprimo alla famiglia e ai suoi affetti più stretti il mio cordoglio. Non è facile ricordare in pochi minuti un uomo dall'alta statura morale, sociale e politica quale è stato Epifani. Voglio però iniziare da alcune sue parole risalenti a quindici anni fa, quando era segretario generale della CGIL, ma ancora profondamente attuali; parole che Epifani usò per rivendicare il ruolo e l'importanza del suo sindacato nel contesto sociale, politico e storico dell'epoca e che credo riassumano perfettamente la missione che egli ha portato avanti durante tutta la sua carriera, prima in Corso d'Italia e poi in Parlamento, come dimostra la presenza in Piazza Santi Apostoli, a Roma, al fianco dei lavoratori della Whirlpool pochi giorni fa, prima della sua scomparsa. «Riprogettare il Paese» scrisse «vuol dire proprio questo: saper aggredire i nodi di fondo di un modello produttivo e sociale che ha generato più disuguaglianze, più povertà, più solitudine; indicare la necessità di definire una proposta e un progetto per la sua ricostruzione, per la sua rinascita civile e morale, partendo (...) dalla centralità del valore del sociale del lavoro»; disuguaglianze, povertà e solitudine che egli aveva toccato con mano quando, da adolescente, dopo esser tornato a Roma da Milano, andava a fare ripetizioni ai bambini delle famiglie più svantaggiate e ad assistere gli anziani. Anche per questo, nel percorso di ricostruzione che l'Italia si appresta a fare per uscire dalla pandemia, la saggezza, la coerenza, la propensione al dialogo e al confronto, l'equilibrio e la determinazione di Guglielmo Epifani, che in prima persona ho avuto modo di apprezzare, sarebbero stati un bene preziosissimo per tutti noi. Più volte, nell'anno e mezzo in cui ho ricoperto l'incarico di Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ho avuto l'opportunità e la fortuna di confrontarmi con lui sia in pubblico, sia in privato. L'esigenza di garantire un lavoro più dignitoso, soprattutto per le nuove generazioni e per le donne, quella di sostenere il lavoro nei settori a bassa produttività, la grande attenzione alle crisi aziendali e occupazionali, nonché la necessità di investire in ricerca e formazione erano temi ricorrenti durante i nostri colloqui. Tra i numerosi obiettivi che condividevamo, c'era anche quello prioritario di assicurare a tutti i lavoratori una maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro; questo perché a ricordarlo oggi è stata anche la senatrice Malpezzi - come ha detto Epifani in uno dei suoi ultimi interventi in Aula alla Camera, tutto dipende dalla salute e dalla sicurezza delle persone: lo stato del presente, la possibilità di programmare il futuro, gli interessi economici, la propria dignità, la propria libertà, il proprio lavoro, il sistema degli affetti di relazione. «Grandezza significa: dare direzione. Nessun fiume è di per sé grande e ricco: è il fatto di accogliere e di convogliare in sé tanti affluenti ciò che lo rende tale». La grandezza di Guglielmo Epifani, un *leader* colto, pragmatico e inclusivo, è stata quella di non cambiare mai strada andando sempre incontro ai lavoratori e ai loro diritti. Sta a noi continuare a seguirla onorandone quotidianamente la memoria. Signor Presidente, onorevoli senatori, voglio aggiungere le mie parole in senso di cordoglio, a nome del Governo italiano, a seguito di questa scomparsa che lascia un vuoto incolmabile. Ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi e la loro misura dà anche il senso della personalità con cui abbiamo a che fare, una personalità evidentemente di parte, con un'idea chiara e netta, ma sempre pronta a dialogare con tutti e interprete del mandato costituzionale. La nostra Costituzione ci richiede di assumere e svolgere le nostre funzioni con disciplina ed onore e credo che la figura di Guglielmo Epifani abbia saputo rappresentare a testa alta e con assoluta qualità esattamente queste funzioni. Guglielmo era un grande intellettuale, ma al tempo stesso un uomo pragmatico e popolare. Guglielmo era al tempo stesso una persona ferma sui principi, rigorosissima sulle grandi questioni, ma sempre attenta alle opinioni degli altri, sempre accorta, garbata, curiosa di comprendere e di capire anche l'opinione di chi la pensava in maniera diversa. sono il lavoro e la difesa del diritto al lavoro come matrice essenziale della sua vita. Credo che non sia stato un caso, ma forse una volontà di Dio, quella di vederlo protagonista per l'ultima volta a pochi giorni dalla sua scomparsa proprio in una piazza, a fianco ai lavoratori della Whirlpool. Lui è stato per l'intera esistenza a fianco a chi si batte per difendere il lavoro come tratto essenziale dell'identità e della vita di ciascuno. Era socialista, come spesso è stato richiamato in queste settimane. A me piace dire che la sua idea di socialismo era intrisa di umanesimo: un socialismo inteso come tentativo quotidiano di costruire una realtà diversa, in cui a ciascuno potesse essere offerta un'opportunità, in cui nessuno venisse lasciato indietro e in cui dappertutto, in ogni angolo del mondo, si potesse combattere per allargare i diritti, per dare più diritti a tutti. In conclusione, voglio ringraziarvi per le parole che avete voluto usare, senza differenze di colori, nel ricordo di questa personalità. Aggiungo chiaramente il cordoglio del Governo e l'impegno a tenere viva quella lezione: una lezione di natura costituzionale, che credo debba coinvolgerci tutti nelle prossime difficili e complicate sfide che il Paese dovrà affrontare.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento

rappresentante del Governo, senatrici e senatori, il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire si pone in diretta successione, ma in netta e profonda discontinuità, con una serie di provvedimenti che lo hanno preceduto e che hanno imposto misure restrittive per contenere l'epidemia da Covid-19. Questo decreto è l'ultimo tassello del mosaico normativo che ha caratterizzato la vita del Paese nell'ultimo anno. Non possiamo non esprimere una soddisfazione, chiaramente mitigata dagli effetti del Covid, che ci sono ancora - ci mancherebbe - perché il virus non è sparito e produce ancora sofferenza e morte. È chiaro, però, che negli ultimi mesi abbiamo avvertito un deciso cambio di passo con il Governo Draghi, attraverso scelte chiare e nette, nette, come possiamo vedere alla luce di una campagna vaccinale finalmente vigorosa: oltre 42 milioni di somministrazioni, 2.700 punti vaccinali - altro che "le Primule", di cui si parlava tanto, da 8,5 milioni di euro, su cui bisognerà poi fare chiarezza nelle prossime settimane - 14 milioni di cittadini vaccinati con due dosi, con un miglioramento complessivo radicale

essere, attesa da tutte le attività che hanno più sofferto le pesantissime conseguenze della pandemia. Il sistema è stato difeso negli ultimi mesi con dei ristori, necessari sicuramente in parte insufficienti, ma non c'erano alternative alle limitazioni imposte, perché doveva prevalere la cura della sicurezza pubblica in termini di salute, oltre alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per arrivare a questo percorso virtuoso. Quattro mesi fa sembrava impossibile ipotizzare o tracciare una situazione di questo tipo. Come forza politica siamo stati sostenitori decisivi di un cambio di passo, in quel momento avversati, considerati in qualche modo gli sfasciacarrozze della situazione, mentre i risultati testimoniano come ci fosse bisogno veramente di un cambiamento, di una nuova iniziativa di Governo e quanto il Governo attuale sta facendo va nella direzione da noi auspicata. Si tratta di un cambio di passo anche dal punto di vista delle modalità di lavoro:

come sta facendo il Senato e come è stato fatto alla Camera nelle settimane precedenti - introdurre modifiche e ridare slancio alla partecipazione parlamentare come punto cruciale e nevralgico della vita della nostra democrazia. Considerando l'evoluzione positiva del quadro epidemiologico, il decreto-legge prevede una serie di misure che ormai conosciamo e che sono patrimonio comune dei nostri cittadini, che hanno visto un progressivo riaprire delle attività, un miglioramento delle possibilità di mobilità: il 7 giugno il coprifuoco è stato spostato alle ore 24, e dal prossimo 21 giugno cesserà; con il passaggio di dodici Regioni nella colorazione bianca, nel loro territorio si ripristina una totale libertà di movimento. Sono state riaperte le scuole e c'è stata la riapertura dei ristoranti, prima all'aperto e ora anche al chiuso: attività che hanno sofferto pesantemente, ma che ora vedono vedono un po' di luce in fondo al tunnel. Il decreto-legge in discussione prevede inoltre la progressiva di apertura dei musei, delle palestre, delle piscine e di tutti i luoghi di cultura e di socialità. Dal 1° luglio riapriranno anche i centri termali, i parchi tematici e sono già tornati ad essere organizzati cerimonie, matrimoni ed eventi: un settore della società e dell'economia che spesso non è stato considerato adeguatamente; il *wedding* ha perso tantissimo e c'è stata sofferenza di tanti imprenditori di quel settore, magari non sotto i riflettori come altre attività, che hanno pagato un duro prezzo ma ora vedono anche loro una nuova luce in fondo al tunnel. Altro aspetto importante è il *green pass* vaccinale. vaccinale. Il Governo italiano ha anticipato il disegno europeo del *green pass* prevedendone la validità fin dai quindici giorni successivi alla somministrazione della prima dose e per i successivi il Governo Draghi ha dimostrato tempismo e il Parlamento ha dimostrato la capacità di recepire le indicazioni del Governo. Che ci siano dei passi avanti lo testimoniano anche dei dati recenti dell'osservatorio dei conti pubblici di Cottarelli, che hanno evidenziato che il il rilassamento delle restrizioni, che il decreto del 22 aprile ha determinato, ha portato a un miglioramento della mobilità. Addirittura, i dati per quanto riguarda gli spostamenti in macchina e con i mezzi pubblici sono superiori al livello del 13 gennaio 2020, in periodo *pre* Covid. Ciò significa che il Paese sente in maniera determinata un clima di ripartenza, ed è questo che noi dobbiamo cercare di accompagnare,

Ci deve essere ancora attenzione, ma fa parte della cultura degli italiani, perché questo anno non sarà dimenticato facilmente. Noi crediamo che questo sia un provvedimento costruito nel solco del rischio calcolato, che qualche mese fa fece storcere il naso a qualcuno, ma in realtà conteneva un'indicazione chiara che il Governo voleva dare: ripartire con dei piccoli passi. Ma se quella ripartenza è stata possibile e i piccoli passi ora stanno diventando più grandi, lo dobbiamo all'attenzione del Governo e del Presidente del Consiglio, che noi sosteniamo con convinzione non solo alla luce di ciò che sta facendo nel campo della lotta alla pandemia, visti i risultati sotto gli occhi di tutti: lo sosteniamo con convinzione in una fase di ricollocazione nel nostro Paese al livello che merita. Abbiamo visto il successo che c'è stato anche nel G7 recente; c'entra poco magari con la pandemia, ma sicuramente la ripresa dei Paesi dopo la pandemia è stata la base di quell'incontro in Cornovaglia in cui il nostro *Premier* ha rappresentato l'Italia nel modo migliore e ha ricollocato il nostro Paese nella chiarezza delle alleanze che storicamente lo hanno caratterizzato (l'atlantismo, l'europeismo), qualcosa che per noi è fondamentale e lo deve essere per questo Parlamento. Dispiace che, mentre il nostro Presidente era impegnato in quello sforzo diplomatico e politico, qualcuno ha preferito incontrare l'ambasciatore della Cina, Paese che noi rispettiamo profondamente perché abbiamo

economiche ed anche politiche, ma che sicuramente non fa parte del nostro modo di intendere, soprattutto per quanto riguarda i diritti umani, i rapporti politici e la quotidianità della vita. Ben venga l'impegno del nostro Presidente, che continuiamo a sostenere con convinzione. Il Parlamento ha il dovere - come ha fatto già per questo decreto - di lavorare al fianco del Governo, garantendo la conversione dei decreti-legge e il miglioramento degli stessi, dando al Paese lo slancio per uscire da una crisi difficile che nei prossimi mesi mostrerà ancora il segno. Con questi provvedimenti e con una tale questa determinazione, però, si consentirà al Paese di rivedere la luce.

Il Governo Conte nel 2020 ha emanato 35 decreti e ha posto 10 volte la fiducia.

perché, con una maggioranza così enorme, porre la questione di fiducia è un fatto istituzionalmente inconcepibile e incomprensibile. in più questa ennesima posizione fiducia nella prima tornata della valutazione parlamentare della conversione del decreto, e cioè alla Camera, innova anche una sorta di autoriforma delle istituzioni, che ci ha visto colpevolissimamente inclini ad annullare un ramo del Parlamento

Con questo provvedimento abbiamo innovato ulteriormente e abbiamo pensato, pur avendo a disposizione un'ipertrofia di maggioranza, di

su una sorta di atto dovuto che deve ragionevolmente e velocemente integrare un vuoto normativo: lo facciamo sull'atto più importante che gli italiani aspettano da oltre un anno, cioè da oltre quindici mesi, che prevede come, quando e perché riaprire

dell'attività del Governo che agisce in totale noncuranza del necessario confronto nei livelli istituzionali costituzionalmente preposti

Continua la prassi delle decisioni assolutamente incomprensibili, che non trovano un logico riscontro e che la gente non capisce.

di Asso Intrattenimento: un comparto assolutamente importante che attiene al mondo - per così dire - della notte, delle sale da ballo, delle discoteche, dei locali dove ci si intrattiene

sotto i colpi dei provvedimenti del Governo che, latitante sul versante del contenimento sanitario della pandemia, si è trovato costretto a dover agire sul versante della limitazione delle libertà individuali e di impresa. Questo Questo mondo oggi non capisce che cosa deve fare. Nel decreto-legge in esame non sono contenuti i chiarimenti necessari; i Comuni agiscono in totale libertà di giudizio e inevitabilmente i sindaci devono colmare le lacune dei provvedimenti del Governo che non parlano chiaro ed equiparano una discoteca o un locale

a dir poco a singhiozzo, una non ripartenza. Oggi siamo di fronte all'ennesimo provvedimento non condiviso da gran parte degli operatori del nostro Paese.

Il ministro Speranza ha pensato bene di allontanarsi, perché evidentemente il provvedimento che attiene alla ripartenza non è roba sua; lascia il Ministero degnamente rappresentato dal collega Sileri e vorrei dire che non sentiamo la mancanza del ministro Speranza, se non a livello istituzionale. Venuto in Aula correttamente e giustamente per raccontarci il suo dolore per la perdita del del compianto Guglielmo Epifani, poteva almeno avere l'accortezza di trattenersi per un caffè con noi, per trattare un provvedimento che l'Italia aspetta da oltre un anno. Comunque, tant'è. Il provvedimento Il provvedimento ci desta preoccupazione ulteriore sul versante del tracciamento. Collega Sileri, noi abbiamo perso il tracciamento nel momento in cui la pandemia ci ha superato,

Se, anche con i numeri attuali, non riusciamo a ripristinare il tracciamento, siamo fottuti e mi scuso con la Presidenza per aver usato un termine forte, ma

per definizione deve essere personale, individuale; deve essere un certificato, che, incredibilmente, ci dà la possibilità nella speranza di qualcuno, che io credo sia poco normale - di entrare al ristorante, di andare a teatro, di giocare una partita a calcetto. Siamo veramente

è un provvedimento che segna finalmente una inversione di tendenza e lascia finalmente intravedere una luce in fondo al tunnel; certo, una luce ancora non definitiva, ma una luce. Lo aspettavamo noi e lo aspettavano sicuramente ancora di più gli italiani, tante famiglie, tanti lavoratori, tanti ragazzi che hanno atteso finalmente un cambio di passo. Con questo provvedimento delineiamo gli ultimi tornanti di una salita che, però, non è ancora conclusa e che, quindi, va affrontata, ancora nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, con prudenza e rigore, proprio in questa fase più necessaria che mai. Si tratta di un atto che si inserisce in un quadro di interventi molto complessi e articolati, che negli ultimi mesi ci hanno aiutato a fronteggiare l'emergenza e che, dal punto di vista anche di una cornice dell'ordinamento, sostanzialmente sono stati definiti da provvedimenti, anche molto articolati e diversi tra loro, che però in quest'Aula tutti ben conosciamo e sui quali è inutile ritornare. ritornare. In questo contesto è forse più utile ricordare che, a un certo punto, con una scelta anche consapevole, rispetto alla quale il Partito Democratico è stato deciso, abbiamo deciso di abbandonare lo strumento dei DPCM. DPCM. L'abbiamo ritenuta una scelta qualificante in nome del coinvolgimento del Parlamento in una fase in cui - come ricordiamo tutti - nonostante scelte fatte, servivano però tempi molto rapidi nelle decisioni. Questo decreto riconosce lo stato di emergenza al 31 luglio e definisce, al contempo, un percorso di riapertura delle attività, tali da conciliare l'attenzione verso l'evolversi del virus con la necessità però di riprendere attività economiche, sociali e culturali che durante questo anno e mezzo sono state interrotte. In tutti questi mesi il Partito Democratico, nelle aule parlamentari ma anche e soprattutto nella sua azione di Governo, ha cercato di tenere sempre fermo il principio, per noi indispensabile, ieri come oggi, di precauzione e prudenza. Ha sempre difeso l'idea che la soluzione dell'emergenza sanitaria non potesse venire se non dalla scienza e dagli strumenti, a partire ovviamente dal vaccino dalle competenze straordinarie di medici e di ricercatori ai quali era doveroso prestare attenzione. *(Applausi)*. Lo voglio dire con forza: lo era ieri, lo è oggi e lo sarà domani, anche fuori dall'emergenza. Lo abbiamo fatto nella consapevolezza che una pandemia di questo tipo richiedeva che la politica facesse non un passo indietro, ma almeno un passo di lato, trovando il modo di dialogare in maniera rigorosa, accorta e decisa con tutta la comunità scientifica. E così abbiamo fatto. Non è stato sempre facile, ma oggi forse, finalmente, seppur sommessamente, guardando alle scelte passate, possiamo dire che è stato giusto fare tutto questo: fare ogni sforzo per non contrapporre diritti contro diritti, cercando di trovare sempre un equilibrio delicato, certamente difficile e faticoso, ma necessario, tra diritto universale alla salute e tutela di tutte le altre libertà personali. Questo anche per ribadire, ancora una volta, che lo stato di emergenza non è mai stata una delega in bianco al Governo, come pure qualcuno ha provato a dire. È stato, invece, uno strumento che ci ha dato la possibilità di agire, ma non ha concesso mai alcun automatismo. Prova ne è il fatto che oggi, proprio prorogando l'emergenza, il decreto conferma, invece, una tendenza diversa: estendere riaperture e nuovo inizio. permesso una gradualità delle aperture, che oggi ci fa assistere al rallentamento costante dei contagi, dovuto in primo luogo al successo della campagna vaccinale, ma anche alle norme che abbiamo messo in campo per definire il calendario del progressivo allentamento delle restrizioni e delle limitazioni agli spostamenti.

questo documento servirà ad attestare l'effettuazione della vaccinazione anti-Covid; sarà fondamentale e consentirà l'uscita temporanea da alcune strutture residenziali e l'assistenza in sala d'attesa anche per gli accompagnatori dei pazienti affetti da Covid. Queste norme, oltre a giustificare la forma legislativa del decreto-legge, dimostrano un lavoro parlamentare efficace e rappresentano un passo in avanti considerevole nello sforzo che il nostro Paese, il Governo e il Parlamento hanno compiuto e stanno ancora compiendo per affrontare l'emergenza sanitaria.

chi ha subito gravi perdite nelle proprie attività o addirittura il proprio lavoro. Tra questi, voglio ovviamente ricordare donne e giovani che - come sappiamo - stanno pagando il prezzo più alto della crisi. Per tutto questo, forte è stato l'impegno che abbiamo messo in campo nei mesi passati e soprattutto in alcuni momenti, anche per le difficoltà di una presenza fisica nell'attività parlamentare. Questo impegno dovrà continuare con altrettanta forza nei mesi che ci attendono, che speriamo saranno migliori dal punto di vista sanitario, ma che che potranno essere più difficili per l'emergenza sociale ed economica che ci attende. Siamo entrati in questa pandemia con forti disuguaglianze tra livelli di inclusione, l'abbiamo attraversata con differenze tra chi è stato più garantito e chi meno e oggi ne usciamo con quei divari che purtroppo si sono allargati e approfonditi. È pertanto indispensabile - come ci ripete spesso il Presidente del Consiglio - lavorare per un'inclusione di tutte e tutti, al fine di creare le migliori condizioni per lo sviluppo del Paese. Sanità territoriale, scuola, lavoro e *welfare*: è questa la strategia per il futuro che non si limiti ai prossimi anni, ma progetti in maniera coraggiosa

(sia essa di genere, di generazione, di territorio e di settori economici e sociali). Il nostro partito partecipa con convinzione a questo Governo e ne sostiene la sua agenda ambiziosa, anche collaborando con forze politiche eterogenee, perché sa quanto sia importante oggi per ripartire e restituire all'Italia la forza per costruire, anche su basi nuove, il proprio futuro. Ce lo chiedono gli italiani, le donne e i giovani che hanno sopportato tanti sacrifici che noi abbiamo il dovere di non sprecare. Il percorso avviato di ritorno alla normalità è la dimostrazione più chiara di quanto tutti noi teniamo alla difesa delle libertà individuali e collettive che soltanto una democrazia compiuta,

le misure dirette all'allentamento di tutte le limitazioni, segna la fase della ripartenza. È quindi un momento

dell'ultimo anno e mezzo, a mio avviso, ci hanno permesso di arrivare a questi risultati.

togliere il coprifuoco e chi lo voleva mantenere, e tutti gli elementi di prudenza che sono stati portati avanti ci permettono oggi di poter finalmente avere un Paese

siamo in una fase diversa, ma io penso che non dobbiamo mai far venir meno i principi di cui parlavo prima, cioè i principi di precauzione e di prudenza.

Il collega di Fratelli d'Italia ha fatto riferimento, per esempio, alla questione del tracciamento. Penso sia una questione che oggi dovremmo affrontare con molta serietà, perché il numero dei contagi è notevolmente ridotto.

ridotti, è possibile a mio avviso avviare una fase che ci permetta, attraverso il tracciamento, di avere un controllo maggiore.

In questo periodo così difficile di crisi pandemica e quindi di emergenza (poi vedremo se

che bisogna investire nel servizio sanitario pubblico; questo è l'altro elemento che ci consegna l'esperienza di questa pandemia. Non basteranno le risorse, che pure sono notevoli, messe all'interno del Piano nazionale di ripresa e di resilienza, ma credo che sarà necessario affrontare fino in fondo, in quest'Aula e nelle sedi competenti...

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, credo che questo vada ricordato come un momento importante, ed è tale perché traccia il confine del passaggio da una situazione emergenziale a una situazione che vuole essere di normalizzazione. Lo accogliamo con grande soddisfazione. Credo di non svelare alcun segreto se dico che, all'interno del Consiglio dei ministri, i partiti del centrodestra sono stati quelli che, per per primi e con maggiore insistenza, hanno chiesto al presidente Draghi e a tutta la compagine governativa di allargare i cordoni delle restrizioni per consentire un graduale ritorno alla normalità. normalità. Questo atteggiamento, questa attività che ha portato a un confronto serrato, molte volte anche ruvido - ma a mio avviso necessario per le finalità che si proponeva

concedere ai cittadini quel senso di responsabilità, quel credito che sicuramente hanno diritto di vantare. D'altra parte, non era possibile aspettare la definitiva uscita dalla pandemia per riaprire le attività commerciali, imprenditoriali e lavorative, che hanno visto in questi anni ipotecare, per necessità, il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti con continui scostamenti di bilancio che sono serviti non a risarcire, ma ad alleviare il più possibile i danni e le sofferenze del settore economico. Leggiamo quotidianamente di attività commerciali e di ristorazione, di bar che chiudono, quindi, probabilmente, secondo il nostro punto di vista, avremmo dovuto iniziare prima ad allentare questa situazione di rigidità nei movimenti e nell'esercizio delle attività commerciali. Siamo comunque soddisfatti del fatto ciò si è verificato. Prendiamo anche atto di un cambiamento, di un'inversione di tendenza: siamo passati dai DPCM - che praticamente mettevano il Parlamento, ma anche il Capo dello Stato, nella posizione di spettatori inermi delle iniziative del Presidente del Consiglio - alla fase dei decreti-legge, che sono sicuramente frutto di un momento emergenziale, ma che fanno partecipare il Parlamento all'*iter* all'*iter* di conversione legislativa e, come in questo caso, danno la possibilità di introdurre ulteriori elementi, dal nostro punto di vista anche migliorativi. Dobbiamo continuare su questa strada. Il momento emergenziale terminerà il 31 luglio; leggevo questa mattina della possibilità di prorogarlo fino al 31 dicembre. Credo che questo debba essere un atteggiamento preventivo nella speranza che non ce ne sia bisogno, diamo comunque la possibilità al Governo - fino a quella data - di intervenire in maniera tempestiva su eventuali resipiscenze. La pandemia non è completamente sconfitta; sicuramente le percentuali ci dicono che la campagna di vaccinazione e l'educazione a rispettare le misure minime di sicurezza da parte dei cittadini hanno contribuito moltissimo a ridurre quotidianamente il numero delle delle infezioni e hanno praticamente portato alla normalità le situazioni dei nostri ospedali che, per un certo periodo, sono stati al limite del collasso. Questo ci deve far riflettere che non possiamo e non dobbiamo più trovarci in questa situazione. Noi ci auguriamo che le somme destinate al Piano di ripresa e resilienza siano investite adeguatamente, per consentire di ripagare i sacrifici che abbiamo chiesto alle future generazioni con investimenti per la riaccensione dei motori dell'economia, che possa consentire a tutti di avere una prospettiva di lavoro adeguata. Signor Presidente, sicuramente

abbia diritto di essere ribadita dai rappresentanti della maggioranza. È questa una maggioranza istituzionale, fatta nell'interesse del Paese; ogni partito che sostiene questo Governo ha fatto una scelta di campo: ha preferito le ragioni del Paese piuttosto che gli interessi del proprio partito, non guardando i sondaggi e non parlando alla pancia dei cittadini, che in un momento di difficoltà chiaramente hanno il diritto di protestare. Tuttavia, signor Presidente, non è possibile che un ramo del Parlamento - in questo caso, il Senato della Repubblica - abbia una funzione esclusivamente di ratifica del lavoro svolto dalla Camera dei deputati. Questa cosa non è possibile. Lo dico perché, mentre ci accingiamo a convertire questo decreto-legge, alla Camera dei deputati sono in discussione il decreto-legge sostegni-*bis*, il decreto-legge

dare soltanto un tributo di firma a un'attività che altri svolgono, senza coordinamento tra i vari rami del Parlamento, senza che i senatori possano partecipare e intervenire in questo processo di conversione di decreti-legge. Mi auguro che per il futuro ci sia un adeguato bilanciamento e il rispetto delle prerogative legislative del Senato della Repubblica, che non può essere semplice spettatore, né può essere chiamato soltanto a ratificare. La nostra è ancora una Repubblica parlamentare fondata sul bicameralismo perfetto, quindi credo che il Senato abbia le stesse prerogative e gli stessi diritti di affrontare e di intervenire nei processi legislativi.

restrittive, ma avremmo inserito altri elementi. Avevamo proposto emendamenti, che poi abbiamo ritirato, che miravano a prevedere che l'inizio dell'anno scolastico fosse sicuramente in presenza e fosse data la possibilità a chi di competenza di organizzarsi per tempo, per mai più tornare a quello che noi abbiamo vissuto sulla pelle dei nostri giovani, dei nostri figli, che hanno praticamente perso due anni di attività didattica in presenza, alla quale avevano diritto. *(Applausi)*. Ma non abbiamo potuto non abbiamo potuto insistere su questi emendamenti, che - ripeto - per senso di responsabilità abbiamo ritirato. Tutto questo per dire, signor Presidente, che noi ci aspettiamo per il futuro una una pari dignità rispetto alla Camera dei deputati. Non capiamo per quale motivo si debba caricare un ramo del Parlamento in maniera così evidente e pressante, lasciando l'altro ramo a occuparsi dell'ordinaria amministrazione e a ratificare i provvedimenti trasmessi dalla Camera dei deputati. Mi auguro che per il futuro anche la signoria vostra voglia tenere in considerazione questa

sostanzialmente la sintesi di due decreti precedenti che, in continuità con altri provvedimenti adottati dall'attuale Governo, ma anche dal Governo precedente, sono volti a gestire la situazione creatasi dopo la pandemia.

Questo, evidentemente, è stato possibile grazie all'efficacia che la campagna vaccinale ha acquisito con il passare dei giorni, efficacia che è andata via via crescendo, che ci consentirà presumibilmente di arrivare all'immunità di gregge entro il prossimo settembre, condizione evidentemente indispensabile per un rientro nella piena normalità. Per questo rivolgo il mio plauso al generale Figliuolo e ai governatori delle Regioni che si sono fatti trovare pronti per le necessità a cui sono stati richiamati. Merito, però, va anche agli italiani, che con stoicismo, con senso di responsabilità, con quella condivisione dell'obiettivo che ha caratterizzato moltissimi di noi, si sono adeguati alle misure previste e questo ha fatto sì che i numeri dei positivi al contagio si siano ridotti a quella quota residuale che tutti noi conosciamo e che è diventata una costante degli ultimi giorni. Ora l'obiettivo è far ripartire il Paese. La mia esperienza professionale mi fa vedere un rischio davanti a noi, un burrone in cui rischiamo di cadere. So, per aver fatto questo lavoro per tanti anni, che siamo in prossimità della chiusura di un ciclo economico. L'economia procede per cicli, quindi a momenti favorevoli inevitabilmente conseguono movimenti di minor favore secondo me il calo dei mercati del 2020, essendo stato determinato da una causa patologica, non rappresenta la fine del ciclo, ma in realtà non ci consente di dire che siamo usciti da un ciclo economico positivo che dura da più di 10 anni, uno dei più lunghi di tutti i tempi. Questo mi consente di arrivare alla considerazione di cui dicevo prima: secondo me, in questo momento, corriamo il rischio che la fine di un ciclo economico positivo ci lasci impreparati nell'eventualità che si dovesse arrivare ad adottare misure di contrasto e questo è sempre necessario. Se chiedessi a ciascuno dei presenti qual è stata la crisi economica più grave di tutti i tempi, tutti risponderebbero che è stata quella del 1929 e avrebbero ragione, non perché nei suoi termini fondamentali fosse effettivamente così grave, ma perché lo è diventata quando, in ottemperanza al principio di non ingerenza della Federal Reserve, si decise di non andare a turbare il normale andamento dei mercati, si consentì la partenza di un effetto domino che poi, a cascata, portò le conseguenze sui mercati che tutti noi conosciamo, quindi alla crisi economica più grave di tutti i tempi. Le crisi possono essere contrastate, anche in termini molto efficaci, con due misure principalmente. La prima è quella dell'immissione di liquidità sui mercati: nel momento di bisogno, le banche centrali immettono liquidità per sostenere i mercati in difficoltà. L'altra arma a disposizione è la riduzione dei tassi, ma in questo momento tutti i Paesi del mondo stanno immettendo sui mercati una quantità di liquidità che non era stata mai in precedenza prevista come sostegno all'economia. Si parla spesso di piano Marshall, ma quel piano era circoscritto nella sua efficacia territoriale, in quanto riguardava un intero continente, ma non riguardava tutto il mondo come sta accadendo ora, perché tutti i Paesi del mondo hanno adottato misure di contrasto alla crisi prevedendo una quantità di liquidità senza precedenti. È fondamentale, quindi, che per far sì che si possa evitare la conseguenza negativa della fine di un ciclo economico queste misure diventino efficaci, quindi va bene che siano state previste misure di sostegno nel *recovery plan*, ma abbiamo la responsabilità di renderle efficaci sia in termini sostanziali, sia in termini di tempo, perché se non fossimo tempestivi rischieremmo di arrivare tardi e quella evidentemente sarebbe una responsabilità a carico di tutti noi. Per fare in modo che le misure diventino efficaci servono le riforme e le semplificazioni.

L'altro elemento è la riduzione dei tassi. Esclusa la Federal Reserve, che ha un minimo di margine in tal senso, in quasi tutti i Paesi evoluti i tassi sono ai minimi storici, sono addirittura negativi i tassi interbancari, tanto che la liquidità è diventata un costo e alcune banche sono arrivate a chiudere i conti correnti con giacenze molto elevate, quindi evidentemente questa non è una possibilità nella nostra disponibilità. il decreto in esame, a mio avviso, è molto importante perché, se pur non perfetto, come qualche collega ha anche evidenziato, è comunque un passo nella giusta direzione,

dei limiti e il progressivo superamento degli stessi in termini di mobilità e di trasferimenti, nonché la riduzione e poi, come chiesto anche da noi, la soppressione dei limiti agli orari, la limitazione e poi la soppressione dei limiti alla convivialità, con l'eliminazione delle restrizioni che attualmente riguardano il settore della ristorazione. consentirà, non solo un pieno recupero della socialità delle persone, ma darà anche un sostanziale aiuto alla nostra economia, come dicevo prima. prima. In queste situazioni è infatti evidente che non si può ragionare per compartimenti stagni, per cui inevitabilmente quello che ha conseguenze in un settore lo ha anche in tutti gli altri. La limitazione delle restrizioni sarà dunque un aiuto sostanziale anche alla nostra economia: non dimentichiamoci che il miglior ristoro saranno le riaperture. Erano fondamentali i ristori nel momento di difficoltà ed è chiaro che non si poteva non sostenere chi non aveva autosufficienza economica, ma non dimentichiamoci mai che il miglior ristoro saranno le riaperture, sarà la ripartenza ripartenza che è necessaria perché la Nazione è allo stremo. Quando un Paese come il nostro è così in difficoltà, diventa il momento della responsabilità. attuale non è il momento della polemica, non può essere il momento della critica sterile. Ben vengano le critiche, quando finalizzate al miglioramento dell'azione di Governo nei confronti di chi ne ha la responsabilità in quel momento, ma le critiche sterili mai servono a qualcosa e, in un momento di grande difficoltà come l'attuale, rischiano di fare danni. dicevo, questo è il momento della responsabilità politica che abbiamo in quanto amministratori, ma anche responsabilità personale, perché ciascuno di noi, secondo me, dovrebbe fare quanto in proprio potere per aiutare gli altri. Nel momento di difficoltà si tende la mano, si cerca di aiutare come e quando è possibile. A tal riguardo voglio riferire di un episodio personale che mi è successo tre settimane fa. Casualmente ho letto su Facebook una serie di insulti rivolti a tutti i politici. Potevo girarmi dall'altra parte e andare oltre, ma non l'ho fatto perché, anziché essere indirizzati ad una precisa parte politica, come avviene di solito, erano generici, rivolti a tutti noi. Ho deciso di approfondire,

La sera stessa coinvolgo il sottosegretario Nisini; la settimana dopo quella persona e tutti i suoi colleghi hanno incassato la cassa integrazione, perché nel momento di difficoltà la Lega c'è. *(Applausi)*. È lì che dobbiamo dimostrare di essere presenti e noi lo dimostreremo anche nei prossimi tre mesi, raccogliendo le firme per il *referendum,* occasione durante la quale ci sarà un confronto diretto tra tutti noi e gli italiani. Visto che il tempo a mia disposizione purtroppo è quasi finito, chiudo dicendo che sappiamo che questo provvedimento non è perfetto, ma sappiamo altrettanto bene che il meglio è nemico del bene e che la volontà di migliorare per forza delle buone idee spesso le ha rovinate e rese inefficaci. Quindi,

signor Sottosegretario, colleghe senatrici e colleghi senatori, da qualche giorno milioni di italiani vivono in zona bianca e possono fruire dell'allentamento di molte delle restrizioni fino ad ora imposte dalla lotta al coronavirus. Ciò è merito sicuramente del comportamento di tutti gli italiani, ma è soprattutto la conseguenza dei provvedimenti adottati e l'effetto della linea rigorosa mantenuta dai Governi che hanno affrontato questa pandemia, che non sono mai corsi dietro ai ripetuti proclami di quanti hanno cercato, spesso irragionevolmente, di precorrere i tempi. che, invece, sono dettati dai risultati che si raggiungono gradualmente con le misure giuste, come evidenziato dal calo dei contagi, dalla riduzione dei ricoveri in terapia intensiva e dalla diminuzione dei decessi di queste ultime settimane. Le riaperture dovranno avvenire nel rispetto di obblighi che rimangono fermi (distanziamento fisico, indossare le mascherine, lavare frequentemente le mani), perché la lotta al virus non è ancora conclusa, e ce lo ricorda purtroppo quanto sta accadendo in Gran Bretagna, dove, per il rapido diffondersi della variante Delta, quella indiana, divenuta dominante nel Paese, il *premier* Johnson è stato costretto a differire il giorno tanto atteso delle riaperture. Uno studio pubblicato nei giorni scorsi su «The Lancet», una prestigiosa rivista scientifica medica, ha dimostrato che la variante Delta riduce moderatamente l'efficacia dei vaccini.

Quindi la prosecuzione della campagna vaccinale risulta cruciale per la ripartenza. L'effetto delle vaccinazioni ha permesso di mettere in protezione una larga parte della popolazione sopra i settant'anni. Ciò ha fatto sì che da maggio la circolazione del virus si sia maggiormente diffusa nelle fasce di età più giovani. La sfida ora non è solo vaccinare queste persone più giovani, ma anche convincere quella parte di popolazione che, in ogni fascia di età, risulta ancora indecisa. In tale sfida risulta cruciale il ruolo del medico di medicina generale, primo attore delle cure primarie, che conosce i propri pazienti con i quali ha instaurato uno stretto rapporto fiduciario. L'alleanza medico di medicina generale e paziente si rivela decisiva come sempre. La medicina del prossimo futuro, quella disegnata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, passerà anche dalla implementazione della medicina del territorio e delle cure primarie. Un altro patto che si deve mantenere ben saldo è quello tra sanità pubblica e cittadini: la sanità pubblica offre gratuitamente la vaccinazione indicando gli obiettivi da raggiungere in modo che il cittadino possa decidere di accettare l'offerta vaccinale avendo chiari il beneficio da trarre e il rischio connesso, perché la decisione di sottoporsi al trattamento sanitario avviene dietro consenso informato e formato bene. A questo proposito, mi preme dire che una giusta e corretta informazione dovrebbe associarsi alla rinuncia del protagonismo, specie da parte di quanti non sono addetti ai lavori *(Applausi)*, segnatamente in relazione a specifici argomenti di salute e medicina, argomenti per i quali le opinioni devono formarsi sulla base di documentate evidenze scientifiche. È giusto pertanto che siano poche le voci a parlare: in questi casi, quelle delle autorità preposte alla regolazione e alla farmacovigilanza, con buona pace dei vari commentatori che ogni giorno si sperticano su quotidiani e *media* per dire la propria. L'infodemia, ossia l'epidemia di informazioni, rischia di ingenerare nella popolazione soltanto confusione ed allarmismo, ed è condivisibile l'opinione di quanti affermano che decidere se accettare o meno l'offerta vaccinale non significa diritto di scelta del tipo di vaccino da parte del paziente. Prendo spunto dalle parole di Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale dell'ordine dei medici, quando ricorda che i vaccini non sono giocattoli. Come tutti i farmaci, anche i vaccini hanno effetti collaterali, motivo per il quale si prevede una prescrizione del medico e, quindi, un'assunzione di responsabilità di quest'ultimo sia in sede civile che penale. Il ragionamento riguardo a quale vaccino debba essere somministrato spetta al medico, anche se il cittadino può decidere se accettare o meno la scelta del medico. Oggi non è il momento di accampare meriti, di rivendicare primogenitura. Come più volte detto in quest'Aula, è più che mai il momento di lavorare tutti insieme per uscire dalla crisi e porre solide basi per una pronta ripartenza, impegnandosi per poter effettuare campagne vaccinali di massa anche nei Paesi meno capienti finanziariamente. Come giustamente detto, il vaccino è bene comune e, come tale, al di là del giusto riconoscimento per l'impegno in ricerca, deve essere gratuito e non assoggettato a logiche di mercato. Per i predetti motivi possiamo essere fiduciosi nella graduale ripresa delle attività economiche e sociali e per questo motivo il Gruppo MoVimento 5 Stelle voterà a favore del provvedimento oggi in discussione.

il lasciapassare che ci proponete, tra le altre cose, in questo decreto è politicamente discutibile, arbitrario, discriminatorio e, forse, anticostituzionale, ma soprattutto è zeppo di contraddizioni e controsensi. Insomma, vi somiglia. Riepilogando, un vaccino non obbligatorio è uno dei presupposti per un lasciapassare. Ripeto: il vaccino non è obbligatorio. Ciò già basterebbe per chiudere la discussione, ma andiamo avanti. Il vaccino non obbligatorio è giustamente anche gratuito, ma se è gratuito il vaccino perché bisogna pagare per le altre due opzioni del lasciapassare stesso (tamponi e *test*)? Ho capito che il manovratore non va disturbato e che i vaccini sono il vostro mantra, ma così è discriminatorio. Agite sulla disponibilità economica delle famiglie. Chi non si fa gratuitamente il vaccino non obbligatorio deve pagare per tamponi e *test* al fine di ottenere il *pass*, così da spingere a farsi il vaccino. Voi state spingendo le persone a essere cavie e a essere gregge, più che l'immunità di gregge. Il vaccino, però, non sempre vi fa dormire sonni tranquilli. A parte la gente che muore dopo aver fatto i vaccini, ci sono pure quelli che hanno fatto il vaccino, hanno fatto il richiamo, vanno in palestra e, convinti di essere a posto, infettano perché ci sono le varianti. pure quelli che fanno il vaccino e non sviluppano gli anticorpi. A loro date il *pass*, ma seguendo il vostro criterio logico state dando la patente di untori patentati e di untori a norma di legge infatti, siete costretti a parlare di terza dose. Non è dato sapere su quali basi scientifiche, però è così. Ci sono ragazzi che si stanno rovinando solo perché gli avete messo in testa che senza vaccino non sono liberi e lo fate attraverso un'informazione anche telecomandata: la RAI da tv pubblica è diventata tv di Stato. L'altra sera Vespa ha fatto un vergognoso processo a Gianni Rivera, colpevole di avere detto che non si vaccina e, siccome il vaccino non è obbligatorio, lo può dire, come lo può fare. Di contro, Bruno Vespa non può fare bullismo televisivo. Quindi, dico no al vostro lasciapassare. Per essere liberi abbiamo la Costituzione. Prima di passare al voto, permettetemi di esprimere al senatore Fede le congratulazioni mie personali e di tutta l'Assemblea

il presidente Pesco, noi vogliamo denunciare l'immobilismo della maggioranza, che è in confusione e sta paralizzando il Parlamento. Su questo provvedimento debbo dire che siamo

in queste settimane ci siamo completamente bloccati su un decreto-legge che non vale poco, perché vale quasi 31 miliardi di euro. In Commissione bilancio vogliamo denunciare che non si riesce ad esaminare questo provvedimento,

Il presidente Pesco non fa che convocare e sconvocare la Commissione, chiaramente a causa di un forte scontro all'interno della maggioranza. Da ieri sera andiamo avanti a suon di rinvii: almeno tre riunioni della Commissione non si sono proprio svolte. Quindi non si sta discutendo nulla nel merito di a un decreto-legge che, come ripeto, vale una legge di bilancio (quasi 31 miliardi di euro).

per domani saremo nella condizione di poter discutere in Assemblea, perché chiaramente noi in Commissione chiederemo di approfondire i 166 emendamenti, per lavorare su tutta una serie di misure che per Fratelli d'Italia sono di fondamentale importanza. Vogliamo solo ribadire, Presidente, che, come abbiamo sempre detto, questa maggioranza così variegata non va da nessuna parte, non sta producendo nulla di costruttivo e, se ancora dovesse servire, oggi ne abbiamo l'ennesima conferma.

il testo del provvedimento al nostro esame è frutto di un'intesa raggiunta in Commissione a larga maggioranza. L'articolato interviene solo nell'ambito dei procedimenti amministrativi, prevedendo l'utilizzo delle modalità telematiche nel caso in cui ciò sia possibile. Gli articoli da 1 a 5 introducono misure di semplificazione in materia di deposito dei contrassegni elettorali, in materia di autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali, in materia di richiesta del certificato di iscrizione nelle liste elettorali, in materia di richiesta e pubblicazione dei certificati del casellario giudiziario e in materia di designazione dei rappresentanti di lista. L'articolo 1 interviene sia sul testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, sia sul testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali in tema di deposito del contrassegno elettorale, prevedendo che lo stesso possa essere depositato *brevi manu* o su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea. L'articolo 2 interviene sull'articolo 14 della legge 21 marzo del 1990, n. 53 in materia di soggetti competenti ad eseguire l'autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali. Rispetto all'elenco previsto dalla normativa vigente, sono inseriti i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali indipendentemente dalla comunicazione della propria disponibilità. In merito agli avvocati che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, si prevede, in un'ottica di trasparenza, che i relativi nominativi siano tempestivamente pubblicati nel sito istituzionale dell'ordine. L'articolo 3 prevede che il certificato di iscrizione nelle liste elettorali riportante i dati anagrafici e il numero di iscrizione alle liste elettorali dell'elettore, necessario per la sottoscrizione a sostegno di liste di candidati per le elezioni politiche, europee e amministrative, di proposte di *referendum* e per iniziative legislative popolari, possa possa essere richiesto in forma digitale, tramite posta elettronica certificata, dal segretario, presidente o rappresentante legale del partito, del movimento politico o da uno dei soggetti promotori attraverso apposita richiesta all'ufficio elettorale, accompagnata da fotocopia di documento d'identità del richiedente. Si prevede, in caso di richiesta tramite PEC, per sottoscrizioni raccolte a favore di liste dei candidati, che l'ufficio elettorale debba rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. Qualora la richiesta tramite posta elettronica certificata dei certificati sia riferita a *referendum* popolare, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di quarantotto ore dalla domanda. I certificati, rilasciati secondo quanto descritto, costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale. La conformità all'originale delle eventuali copie analogiche dei certificati ricevuti in forma digitale è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da proprio delegato con dichiarazione autentica autografa resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. L'articolo 4 interviene sugli obblighi di pubblicazione previsti per i partiti e i movimenti politici. Si prevede che i rappresentanti legali dei partiti o dei movimenti politici o persona da loro delegata possano richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziario dei candidati, candidato sindaco compreso, previo consenso e su delega dell'interessato. L'articolo 5 stabilizza le modalità semplificate di designazione dei rappresentanti di lista già previste dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25 per le consultazioni elettorali indette per l'anno 2021. Si prevede, in sostanza, sia per le elezioni politiche nazionali, sia per le elezioni amministrative, che l'atto di designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali possa avvenire anche mediante posta elettronica certificata entro il giovedì antecedente la votazione. Inoltre, si prevede che le autenticazioni previste in tale ambito dalla normativa vigente non siano necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente dai delegati e i documenti siano trasmessi a mezzo di posta elettronica certificata. L'articolo 6 dispone sull'entrata in vigore del provvedimento.

Signor Presidente, prima di commentare il merito del provvedimento mi si consenta di esprimere due parole relative al metodo di lavoro. Se siamo in Aula con questo provvedimento è perché nella nostra Commissione ci si è dati un modo di operare innovativo, se un'organizzazione puntuale e precisa dei lavori che si tramuta in efficienza e tempestività. non posso esimermi - e lo faccio con piacere - dal ringraziare e complimentarmi con il presidente Parrini perché ci è da guida in 1a Commissione in questa attività che ha già visto nelle settimane precedenti portare a conclusione un provvedimento sempre connesso a questa materia, e oggi porta in Aula l'Atto Senato 2129. Altri provvedimenti sono in cantiere e, utilizzando lo stesso metodo, riusciremo ad arrivarci con tempestività e in modo molto produttivo. Questa è una strada che tracciamo e che riteniamo debba essere seguita perché consente anche di smussare Nel merito, il provvedimento è composto da cinque articoli, tutti legati alla volontà di semplificare una materia molto tecnica e molto particolare come quella delle procedure preelettorali, al

piccole nicchie di burocrazia che creano impedimento. Con l'articolo 1 offriamo, offriamo, in alternativa alla tradizionale consegna dei simboli, dei contrassegni su cartoncino, in carta lucida, in misura da dieci

un atto di modernità che diamo al sistema di presentazione dei simboli. L'articolo 2 permette di semplificare l'autentica delle firme in caso di elezioni e *referendum* rimuovendo

debba comunque comunicare la sua disponibilità al sindaco ad autenticare le firme. Lo diamo per scontato: il consigliere comunale autentica le firme perché ciò

riguarda la semplificazione della richiesta dei certificati elettorali. Quando si tratta di raccogliere le firme - sappiamo che sono numerose per le elezioni politiche, le elezioni regionali o anche i *referendum* - le firme dei sottoscrittori devono essere accompagnate dal certificato elettorale. A differenza di un'elezione amministrativa in cui l'ufficio elettorale di riferimento è uno solo,

di risparmiare tempo e carta e ciò è significativo per permettere un più facile accesso alle procedure democratiche. L'articolo 4, come ricordava bene e con precisione il relatore, va a sanare l'incongruenza presente in una legge esistente che, a fronte a fronte della mancata presentazione da parte dei candidati del certificato del casellario penale, attribuisce una sanzione al partito di riferimento,

La norma è quasi ottocentesca. Per ogni sezione elettorale di ogni Comune chiamato al voto occorre che i delegati di lista consegnino entro le ore 12 del venerdì una dichiarazione con doppia firma autenticata dei rappresentanti di lista designati in quella singola sezione elettorale. Anche in questo caso, semplifichiamo: tutto potrà avvenire con un unico invio tramite PEC entro la mezzanotte di giovedì, consentendo anche agli uffici di svolgere tutte le operazioni amministrative necessarie. Questo, con con l'articolo 5, è il quinto snellimento burocratico e atto di semplificazione che mettiamo in essere. Signor Presidente, concludo credendo di aver fatto una disamina abbastanza completa del nostro provvedimento. Mi si permetta di ringraziare

ovviamente, per ultimo, ma non ultimo, il rappresentante del Governo, che ci ha assistito e guidato nelle difficili spire dei pareri ministeriali. *(Applausi)*.

dà un'ulteriore dimostrazione del buon andamento e della buona prassi che è nata e che prosegue, in modo ottimale nel Parlamento italiano in conseguenza di questa nuova maggioranza, che si è ritrovata intorno a un progetto di unità nazionale che vede Draghi come Presidente del Consiglio. Si tratta infatti di un provvedimento di iniziativa parlamentare e già questo di per sé depone bene. È un fatto

più evidenti volontà di renderle trasparenti, fino al punto che, forse, sarà complicato trovare candidati disponibili a farsi fare la TAC prima di candidarsi anche solo allo scranno di un Comune di pochi abitanti. in questo caso devo dire però che la volontà semplificatoria è assolutamente necessaria per

C'è stata una leale collaborazione, pur partendo da posizioni distinte, e mi congratulo anche con il relatore, senatore Garruti, per le buone pratiche messe in atto insieme a tutti i colleghi, nessuno escluso, compreso lei, presidente Calderoli, che come sempre, con la sua esperienza e capacità di sintesi, ha dato un evidente contributo

il famoso certificato penale, cioè quello che va estratto dal casellario giudiziale e che era

perché, secondo la precedente normativa, avrebbe dovuto richiederlo e depositarlo agli atti il candidato,

si cerca di colmare una lacuna o, per meglio dire, un vero e proprio errore di impostazione, che determinava per tutti i partiti politici (sia ben chiaro, da quelli di centrosinistra fino a quelli di centrodestra, al MoVimento 5 Stelle) una procedura particolarmente difficile, che certamente stimolava

La seconda questione riguarda i rappresentanti di lista ed era la ragione principale per la quale era stato avviato il procedimento legislativo adesso è possibile una semplificazione in base alle tecnologie più moderne, con la possibilità di indicare i rappresentanti di lista per posta elettronica certificata (PEC), una pratica che ormai è divenuta di uso comune, soprattutto per i liberi professionisti o per chi si occupa di pubblica amministrazione, ed era ovvio che dovesse essere introdotta anche per una procedura che non poteva più essere basata su

L'ultima questione che mi sento di sottolineare è quella dei contrassegni elettorali, che adesso possono essere depositati non solo a mano, ma - anch'essi via PEC, in digitale. Questo è un altro aspetto comunque legato a procedure antiche, ormai superate dai tempi e alle quali con questo provvedimento legislativo si tende ad andare incontro. Concludo questo mio intervento in discussione generale per dire che noi legislatori dovremmo sempre avere un approccio volto alla semplificazione delle procedure.

messa in discussione dell'onorabilità di chiunque voglia intraprendere

di impedimenti, appesantimenti e procedimenti che tendono a supporre che chi fa politica debba per forza farla con un secondo fine, magari illegale. Mi auguro che tutto questo lentamente cominci a far parte del passato e di una cultura sbagliata, sbagliata, che tende non ad avvicinare il cittadino, ma ad allontanarlo sempre di più e a ingenerare il sospetto e l'idea che chiunque voglia avvicinarsi alla politica lo faccia per interessi personali, magari neanche legali, e legali, e non che lo faccia invece per cercare di andare incontro alle esigenze della propria comunità del proprio Paese, per migliorare le qualità della vita di ciascuno di noi. Ecco invece la vera nobiltà che dovrebbe riguardare chiunque si avvicini alla politica. Questo provvedimento è soltanto un piccolo gesto, ma ha un suo valore politico. Ho potuto constatare di persona - e perfino il Sottosegretario n'è meravigliato (e mi farebbe piacere poi sentire anche la sua voce) - quanto, per la prima volta all'interno di un'Assemblea così importante quale quella del Senato, ci sia, da parte di formazioni politiche anche così diverse tra loro e con iniziative politiche che lo sono altrettanto, una volontà comune di trovare soluzioni che riguardano tutti, in modo particolare i cittadini italiani. italiani. Grazie a coloro i quali hanno contribuito a questo risultato. Un ringraziamento particolare lo voglio rivolgere al mio caro amico collega Luigi Vitali, che si è tanto impegnato nel comitato ristretto e a cui va il mio personale applauso.

nel giugno del 2014 si svolsero anche in Italia le elezioni europee. Stefano Patuanelli, in qualità - allora - di delegato effettivo per la circoscrizione nord-orientale, mi nominò sub-delegato per tutta la provincia di Modena, abilitandomi alla nomina dei rappresentanti di lista, incarico che avevo già assunto anche nelle amministrative del 2009 e, successivamente, in tutte le tornate elettorali che hanno riguardato il MoVimento 5 Stelle nelle nove Province della Regione Emilia Romagna. Seguire questi adempimenti burocratici che precedono le giornate dedicate al voto mi ha fatto acquisire esperienza. Voglio ricordare con riconoscenza la responsabile dei servizi demografici del Comune di Sassuolo, dottoressa Giancarla Visconti, per l'aiuto e i consigli operativi di cui faccio ancora tesoro. Discutemmo spesso: aveva sempre ragione lei, ma imparai; non riuscivo a credere che, per trasmettere le nomine dei rappresentanti di lista, non si potesse utilizzare una PEC. Oggi, con il provvedimento in esame, ripariamo anche a questa mancanza. Con la firma digitale si evita pure tutta la procedura di autenticazione della sottoscrizione del nominato. È una soddisfazione rilevare che su un tema tanto importante, quanto tecnico si sia riusciti a trovare una convergenza in pochissimo tempo. Sono trascorse poche settimane dal giorno in cui ho depositato il disegno di legge un testo circoscritto, che, durante l'esame in prima lettura in Senato, è stato notevolmente arricchito dal contributo di numerosi colleghi che ne hanno ampliato l'ambito oggettivo di riferimento. *(Applausi)*. Siamo stati bravi ci attendiamo che i colleghi della Camera dei deputati provvedano senza indugio per quanto di loro competenza. Desidero pertanto ringraziare il relatore, senatore Vincenzo Garruti, il presidente Roberto Calderoli, il senatore Luigi Augussori, il senatore Luigi Vitali, il senatore Nazario Pagano e tutti i Gruppi parlamentari che hanno deciso di condividere lo spirito e il contenuto di questa iniziativa legislativa. Ringrazio anche il senatore Dario Parrini, che a suo tempo, alle mie rimostranze perché in altro provvedimento la modifica che oggi si perfeziona in maniera strutturale aveva una scadenza, mi disse di presentare un disegno di legge dedicato e che lo avrebbe sottoscritto. L'ho preso sul serio e oggi siamo qui pronti e decisi. e decisi. La semplificazione amministrativa, la digitalizzazione e il taglio dell'inutile burocrazia non possono e non devono avere colori politici. L'incredibile progresso tecnologico degli ultimi decenni ci consente e impone oggi di sfruttarne tutte le potenzialità, al servizio dei cittadini e delle nostre Istituzioni. il presente disegno di legge, da una modifica inerente la semplificazione delle procedure pre-elettorali riguardanti la nomina dei rappresentanti di lista da parte dei delegati, ha visto un notevole ampliamento del proprio ambito oggettivo di applicazione, fino a ricomprendere anche importanti semplificazioni in merito al deposito dei contrassegni elettorali, che adesso potrà avvenire mediante formato digitale, in formato vettoriale non modificabile o in triplice esemplare in forma cartacea. introduce anche la possibilità per i consiglieri provinciali, comunali e metropolitani di eseguire le autenticazioni delle firme dei presentatori delle liste elettorali senza doverne comunicare la disponibilità. Si prevede inoltre la possibilità di presentare in formato digitale anche il certificato di iscrizione alle liste elettorali e i certificati rilasciati dai casellari giudiziali. Unanime è stata la volontà di giungere alla rapida approvazione del presente disegno di legge, anche in vista delle elezioni amministrative suppletive del prossimo autunno, per le quali, peraltro, erano già state previste alcune semplificazioni, grazie all'approvazione di un mio emendamento all'ultimo decreto sul differimento della tornata elettorale prevista per questa primavera, così come ho specificato poc'anzi. Quello odierno non è un risultato scontato. Fino all'ultimo ci siamo battuti per superare alcune contrarietà espresse dal Ministero, trovando alla fine un buon punto di caduta. Come rappresentanti del popolo che hanno l'onore di sedere negli scranni di questo altissimo consesso, abbiamo il dovere di ascoltare le istanze provenienti dagli amministratori locali. In virtù del principio di sussidiarietà di cui gli enti territoriali sono espressione, le loro istanze sono quelle dei cittadini e, quindi, delle comunità che rappresentano. Pertanto, è nostro dovere esaminarle al fine gli darvi, laddove possibile, concreta attuazione.

che ho deciso di sottoscrivere convintamente, per intervenire sulla responsabilità penale che grava in capo ai sindaci per i reati omissivi impropri. Un'altra istanza che intendo portare presto all'esame di quest'Assemblea riguarda la possibilità di superare i rigidi limiti presenti nel testo unico delle sul conferimento degli incarichi ai dirigenti collocati in aspettativa. Un'altra battaglia concerne inoltre il riconoscimento dei contributi previdenziali agli amministratori locali che, al momento dell'assunzione dell'incarico, non erano iscritti ad alcuna forma previdenziale.

era il 1979 e, nel suo rapporto alle Camere, uno dei maggiori giuristi europei del XX secolo, Massimo Severo Giannini, scriveva che lo Stato non è un amico sicuro e autorevole, ma una creatura ambigua, irragionevole e lontana. Oggi, a distanza di oltre quarant'anni, molto è cambiato e con l'importante intervento normativo che ci apprestiamo a votare facciamo un ulteriore passo in avanti per ridurre questa distanza e rendere lo Stato un amico sicuro e autorevole per i cittadini, ma anche per i nostri enti territoriali. In conclusione, il modello del MoVimento 5 Stelle ha fatto scuola e i partiti possono chiedere prima delle candidature i certificati penali; vedremo i fatti, non ci sono più scuse.

È un testo che, a mio avviso, ha un valore molto alto, perché la sintesi estrema è rendere più semplice la partecipazione del cittadino alla vita democratica e politica del nostro Paese.

imparo, e credo possano essere un metodo di lavoro che insegna la strada da seguire per portare a casa risultati concreti. Molte cose dividono le forze politiche, però in tal caso c'è l'intento di tutti i partiti politici di tentare in tutti i modi di avere tra le proprie fila persone

rallentare la tempistica del procedimento, inserendo piccoli strumenti tecnologici che permettano ad oggi di velocizzare il processo di presentazione delle liste, che sappiamo essere farraginoso e complesso. Si attualizzano inoltre e soprattutto, grazie anche allo strumento della posta elettronica certificata, riusciamo a velocizzare quel processo, che viene equiparato a un altro, come stabilito nell'articolo 5 approvato dalla Commissione, che dà pari dignità al processo tecnologico rispetto a quello fisico, che viene rappresentato. La possibilità di fare da rappresentante di lista con questi due metodi, potendo trasmettere le informazioni alla pubblica amministrazione in questo modo, apre una strada importantissima,

come sottolineava il senatore Pagano, è veramente un bel segnale quando in poche settimane - diciamocelo pure - uno dei due rami del Parlamento riesce

Oggi purtroppo è successo un fatto a mio avviso raccapricciante: su alcuni siti è stato pubblicato un video relativo alla tragedia della funivia del Mottarone, che mi ha fatto pensare molto, moltissimo, perché con esso si incorre in un incubo che le famiglie continueranno a rivivere. Si vede quando la cabina della funivia arriva alla stazione: in quel mentre, si spezza il cavo. Si vedono, fra l'altro, i visi del piccolo Eitan, del padre e di due signore; poi è stato corretto su alcuni siti, perché l'ho preso dall'applicazione Telegram e comunque era già in larghissima diffusione (è stato diffuso su alcune TV a livello nazionale, sono stati oscurati con dei bollini). La mia domanda è questa: fin dove si spinge il diritto di cronaca? È regolare questo, quando spesso, anche su provvedimenti legati agli atti parlamentari, parliamo di *privacy*?

si possono macchiare di eventi criminosi. *(Applausi)*. Con questo video non vi è nessun rispetto per i vivi e per i morti. Chiedo l'attenzione della Presidenza, di sollecitare le commissioni e gli enti preposti, per verificare come sia potuto uscire, su un fatto del genere, con immagini e apparecchiature sequestrate, un video che viola la *privacy*. Non vorrei trovarmi nei panni di quei familiari che per anni vivranno una vita da incubo nel visionare questo video.

Sarà un'occasione per discutere di un problema sul quale non si riesce a influire e a incidere con la dovuta serietà da molti anni a questa parte.

Abbiamo smantellato tutte le strutture che nel tempo avrebbero potuto farsene carico, perché si sono dimostrate progressivamente inadeguate o prive di quelle competenze e di quel supporto legato a personale di fatto in grado di affiancare, sostenere e supportare queste persone. persone. Mi chiedo fino a che punto dobbiamo lasciare che la salute mentale diventi un obiettivo di cronaca e quando, invece, riusciremo a ricordare che è uno degli obiettivi principali della più grande visione del Sistema sanitario nazionale. Di fatto è noto a tutti che gli investimenti interni in salute mentale sono assolutamente scarsi. Sappiamo quanto profondi siano stati la sofferenza e il disagio, anche in tempo di *lockdown*,

Signor Presidente, gentili colleghi, vorrei svolgere una breve riflessione su uno degli aspetti più drammatici e sottaciuti di questa pandemia, in un momento in cui tutta l'attenzione mediatica e della pubblica opinione è rivolta alle vaccinazioni, dimenticando spesso la disperazione che stanno vivendo moltissimi giovani. L'Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato poco tempo fa un fortissimo allarme e i dati sono stati anche confermati recentemente dall'Istat: il suicidio è la seconda causa di morte nei ragazzi tra i diciannove e i ventiquattro anni. La settimana scorsa c'è stato un ulteriore gesto disperato, quello di un giovane diciottenne che ha ingerito del veleno mentre era collegato a distanza con i suoi amici, che lo incitavano a compiere il folle gesto. Nel calcolo di rischi e benefici, in cui ragazzi come Matteo, Paolo, Fabio o Said - per citare alcuni nomi - hanno scelto di porre fine alla propria esistenza, l'ansia e la solitudine generate dall'emergenza epidemiologica, preclusa la possibilità di vivere qualche momento di spensieratezza, hanno preso il sopravvento, annientando ogni speranza di vita. Si tratta di adolescenti o ragazzi isolati, vittime di soprusi o bullismo, privati per lungo tempo del confronto con altre persone oppure di una semplice uscita con gli amici, senza svaghi e senza distrazioni; quindi, la pressione psicologica è aumentata. L'isolamento e l'emarginazione causati dalla pandemia hanno influito in modo determinante sul graduale e inarrestabile peggioramento delle condizioni psichiatriche in cui versano molti giovani. Per questo molti ragazzi hanno scelto di farla finita, arrivando a preferire la morte piuttosto che lottare quotidianamente contro le proprie ansie e paure. I medici pediatrici hanno lanciato l'allarme già da tempo, dichiarando che c'è stato un aumento di suicidi tra i giovani, nell'ultimo periodo, del 30 per cento. Ci si è chiusi in casa, nella propria stanza, vivendo l'inutilità di ogni relazione; ci si è alienati nel mondo dei *tablet* e degli *smartphone* e qualcuno, purtroppo, non ce l'ha fatta. Terminata l'emergenza, però, sarà ancora più difficile per alcuni ritornare alla normalità; occorre quindi stare attenti e vigili, dando la giusta attenzione anche al più piccolo segnale. Moltissimi ragazzi sicuramente non vorranno comunque uscire di casa, perché, al di fuori del contesto domestico, non si sentiranno più al sicuro, mentre noi qui siamo a ragionare sui grandi poteri e su questioni che, a confronto col drammatico aumento dei suicidi, sono di ben minore importanza, marcando ancora di più la differenza tra istituzioni e Paese reale, tra politica e cittadinanza. Occorre assicurare una tutela adeguata ai nuclei familiari, con la predisposizione di un modello socio-economico che permetta di passare più tempo in presenza con i propri figli. figli. Sarà fondamentale investire sugli sportelli di assistenza pedagogica e psicologica nelle scuole, dove fornire un sostegno pubblico gratuito ai ragazzi e alle ragazze con maggiore difficoltà.

in assenza di colpa e di prove di colpevolezza. Una detenzione arbitraria che si protrae, come uno stillicidio, di udienza in udienza; all'ultima, né ai diplomatici italiani, né a quelli europei è stato permesso di assistere. Una detenzione che è, di fatto, una violazione dei diritti umani, per Zaki così come per altre centinaia di "prigionieri di coscienza". Zaki è costretto a dormire a terra, in condizioni disumane, aggravate dalla pandemia; una detenzione che è già una forma di tortura, un modo per annientare una vita, un pensiero, la libertà di ideali e di convinzioni. Una detenzione per spegnere la luce su Zaki, per far calare il silenzio. Noi all'opposto, invece, dobbiamo parlare a voce alta, come torniamo a fare oggi, se vogliamo salvare Zaki e se vogliamo salvare, con la sua vita, i valori di libertà e di democrazia nei quali crediamo, per i quali hanno lottato i nostri Padri costituenti e su cui poggia la nostra Repubblica. Non è vero che smettere di parlarne aiuta Zaki, perché il silenzio può diventare indifferenza e l'indifferenza è complice. Il nostro Senato ha dato prova di grande dimostrazione di forza politica e di forza morale, chiedendo al Governo di attivarsi urgentemente per il conferimento della cittadinanza italiana a Zaki. Zaki. È la nostra mobilitazione, «siamo noi a tenerlo in vita», ha scritto oggi Ilaria Cucchi, e ha ragione. Il nome di Zaki va portato ad ogni tavolo, in ogni confronto internazionale, finché non verrà liberato. È una battaglia simbolo per la credibilità del nostro Paese. Signor Presidente, a guardare il volto di Zaki si vede il volto di Giulio Regeni, perché entrambi rappresentano la stessa generazione di cittadini del mondo, innamorati dell'Italia, dell'Europa, dell'Egitto; innamorati dei diritti, della libertà di potersi battere per le proprie convinzioni. Parlare di Zaki è parlare di Giulio. Chiedere giustizia per Zaki significa chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni, torturato e ucciso a pochi chilometri da dove Zaki è recluso. Presidente, nell'ultimo incontro che hanno avuto, Zaki ha lasciato alla sua fidanzata un cuore intarsiato nel sapone, a sua mamma una chiesa intarsiata nel legno e poi una lettera per la senatrice Segre, per ringraziarla per il suo sostegno; lei, reclusa nei campi di sterminio, a fianco di Zaki, che è al buio da un anno e mezzo. L'augurio che oggi facciamo è che al più presto Zaki possa incontrare Liliana e tutti noi qui in Senato, consegnare di persona la sua lettera, abbracciarla e riabbracciare,

per sollevare l'attenzione sulla circostanza della vaccinazione ai minori. Tutto quello che sta accadendo in questo momento nel nostro Paese si sostanzia in un clima di incertezza, indefinitezza e non rassicurante informazione nei confronti dei genitori e di chi si deve sottoporre a vaccinazione: pensate solo alle evidenti perplessità alle evidenti perplessità che solleva il vaccino AstraZeneca. Di fronte a questo clima, pensare agli *open day* per la vaccinazione dei minori è una cosa evidentemente deprecabile. Il Gruppo Fratelli d'Italia ha depositato un atto di indirizzo, che speriamo possa essere condiviso dall'intera che sottopone la vicenda al comitato etico dell'Istituto superiore di sanità. Infatti, sulla dubbia eticità di una vaccinazione di massa dei minori per proteggere gli adulti,

delle istituzioni con questo atto di indirizzo. Nei prossimi giorni speriamo di poterlo calendarizzare e sottoporre alla discussione dell'Assemblea.

per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di procedura di nomina dei rappresentanti di lista***